Il nostro primo pensiero - sono certo - si rivolge innanzitutto alle famiglie degli uomini e delle donne uccisi in quell'esplosione. Non erano trascorsi neanche due mesi dalla strage di Capaci quando l'Italia si trovò di fronte un secondo attacco terroristico mafioso. Il 19 luglio è un giorno che racchiude in sé dolore, emozioni, pensieri, ricordi, bilanci e promesse che trovano spazio all'ombra dell'ulivo piantato nel luogo in cui quel tremendo boato trascinò con sé la loro vita e sotto il quale oggi si ritroveranno centinaia di ragazze e di ragazzi. Il dolore e lo sconforto confondono e ridisegnano la nozione che abbiamo del tempo: o cinquantasette giorni sembrano interminabili e, al tempo stesso, volati via in un attimo. La quiete di una domenica qualunque d'estate si trasformò in un istante in una ferita che non potremo mai sanare. Non abbiamo dimenticato nulla di quella domenica palermitana, né della vita né nell'esempio degli uomini e delle donne vittime della furia omicida della mafia. Di Paolo Borsellino voglio in questa solenne occasione ricordare soprattutto il sorriso. Era un uomo solare, simpatico, affabile; professionalmente aveva un eccezionale talento, una passione viscerale e una ineguagliabile capacità di superare fatica e delusioni. Sapeva anche dare il giusto consiglio ai colleghi più giovani; me ne ha dati tanti, preziosissimi, quando iniziai a studiare le carte del maxiprocesso. Dopo il 23 maggio 1992 l'espressione di Paolo si trasformò in una maschera di tensione e di dolore. Fu chiamato dalla sua coscienza a raccogliere il lascito pericoloso del suo amico e collega e, sebbene fisicamente e moralmente distrutto per la perdita di Giovanni, ne assunse la pesante eredità con la precisa consapevolezza che presto avrebbe seguito il suo destino. Aveva deciso di continuare e si era buttato senza un attimo di tregua nelle indagini, imponendosi ritmi massacranti con l'ansia di una vera lotta contro il tempo. Borsellino ha saputo, con la fermezza e la dedizione di un uomo innamorato del suo Paese, dare a tutti noi una grande lezione di coerenza e di senso del dovere. Il suo esempio è sopravvissuto all'esplosivo di via D'Amelio, al tempo, alle calunnie, ai pezzi di verità mancanti che ancora affannosamente cerchiamo. Vive. Vive e si rafforza nei gesti di chi ogni giorno si impegna per la legalità e la giustizia, nella voce di quanti non rimangono più in silenzio, nel coraggio che serve per rifiutare compromessi, privilegi e indebite scorciatoie. Nel nome di Borsellino e in quello di tutti i caduti innocenti per mano mafiosa abbiamo in questi venticinque anni ottenuto molti successi nel contrasto alla criminalità organizzata. Abbiamo sconfitto la Cosa nostra violenta, sanguinaria e stragista, ma non ancora quella capace di mutare pelle, di sparire dai radar dell'opinione pubblica e di infiltrarsi a tutti i livelli nella società, nella politica e nella pubblica amministrazione. Non sono mancati momenti nei quali la mafia ha tentato dei colpi di coda, che ne dimostrano più le debolezza che la forza; penso - ad esempio - ai recenti atti di vandalismo inferti alle statue di due grandi uomini dello Stato: Giovanni Falcone e Rosario Livatino. È proprio dinanzi a questi rigurgiti, alle immagini che ci ricordano l'inferno di via D'Amelio e ai corpi dilaniati che dobbiamo rinnovare la promessa di impegnarci per perseguire ideali di verità e giustizia, e per continuare l'opera di contrasto a ogni manifestazione mafiosa, con uno slancio etico che superi ogni indifferenza e rassegnazione e l'alibi del non sapere. C'è ancora molto da fare e, come membri di questa Assemblea rappresentativa, abbiamo il compito di essere all'altezza di una così decisiva sfida per il nostro Paese e per il nostro futuro. In memoria di Paolo Borsellino, Agostino Catalano, Eddie Walter Cosina, Vincenzo Li Muli, Emanuela Loi e Claudio Traina, invito a un minuto di raccoglimento.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti trasmessi dall'Assemblea al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 1.0.1 (testo 4) e i

Esprime parere non ostativo sulle restanti proposte».

che tenta di mistificare il senso stesso dell'emendamento inserendo una pseudocorrezione e dando la possibilità - e vorrei ben vedere - alla Consip di fare gare per l'acquisto dei vaccini monovalenti.

a seguito della formulazione dell'emendamento del relatore 5.0.3000 (testo 2), che tratta l'ipotesi di acquisto di vaccini monocomponente,

sul quale precedentemente la 5a Commissione aveva posto l'articolo 81, perché ritengo risolva un problema molto importante e colmi un buco presente nel comma 2 dell'articolo 1.

L'esonero dell'obbligo della vaccinazione per avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale di cui all'articolo 1, comma 2, non deve comportare inoculazione dello stesso vaccino in forma combinata».

Credo, tuttavia, che sarebbe opportuno avere una relazione tecnica in proposito, che dimostri che l'ipotesi formulata dall'articolo 5 sia effettivamente in grado di superare il problema.

Presidente, credo che lei abbia fotografato in maniera corretta quanto messo in evidenza sia dal senatore Calderoli che dal collega Arrigoni. Il Ministro probabilmente non ha presente l'emendamento o, purtroppo, sta dando un giudizio per partito preso.

il bando di gara va deserto, perché le aziende non hanno interesse a produrre o a chiedere l'autorizzazione per l'immissione in commercio dei vaccini monocomponenti.

Se conosciamo la realtà, il problema è mettere in atto tutte le azioni necessarie - e forse neanche l'emendamento di cui stiamo parlando ci aiuterebbe a sufficienza - affinché le aziende produttrici non costringano il Parlamento a prendere una decisione sulla base dei piani industriali delle aziende stesse. Se queste non hanno interesse a fare il monocomponente, noi almeno diciamo che ne abbiamo bisogno.

Già imporre l'obbligatorietà in virtù di quelli che sono i prodotti che escono dalle case farmaceutiche, ovvero esavalente e tetravalente, ha poco di serio. Ma non dare nemmeno la possibilità a chi dallo stesso decreto-legge viene riconosciuto come non obbligato alla vaccinazione a procedere

dovete avere rispetto a quella che ha reso invece impossibile il voto sull'emendamento 1.19, perché sempre di monovalenti si parla. Quindi, trovate la quadra anche con voi stessi e cercate di rendere quest'Assemblea meno ridicola di quanto già non si sia dimostrata.

Presidente, le dichiarazioni del ministro Lorenzin su questo argomento ci mettono in grande allarme, perché parla sotto il profilo scientifico e afferma che ciò che sta sostenendo è veritiero. Pongo allora una domanda al Ministro, visto che interviene dal punto di vista scientifico.

alterano la velocità di crescita della cellula e delle membrane cellulari, che sono il primo passaggio per la formazione della patologia degenerativa e, conseguentemente, della patologia tumorale. Visto che parla dal punto di vista scientifico, la invito a rispondere e a dire se effettivamente quello che noi sosteniamo e abbiamo appreso dai giornali, cioè che qualche vaccino contiene mercurio e alluminio, non corrisponde alla verità. Presidente, lei o altri ci volete accusare di fare ostruzionismo? No, signor Presidente. Noi vogliamo difendere i nostri figli e i figli di coloro i quali la pensano diversamente da noi. Il Ministro sa - ed è bugiardo

per aver detto delle falsità in giro per il mondo su questo argomento. Noi non vogliamo fare allarmismi, ma vogliamo parlare ai colleghi, che amano i propri figli quanto noi, per fare chiarezza. Vogliamo trasparenza. Vogliamo che questo decreto si blocchi e si creino

Allora, qual è il supporto all'affermazione del ministro Lorenzin, che parla dal punto di vista tecnico e dal punto di vista scientifico, quando ella stessa non ha le relative competenze scientifiche? Noi, infatti, la riconosciamo come Ministro, ma sotto il

accetto questa sua dichiarazione solo se lei mi porta studi scientifici di soggetti che sono stati vaccinati dopo aver avuto la malattia!

che tutti i Gruppi abbiano richiesto il monocomponente avrà una sua spiegazione logica: oppure è semplicemente per fare uno *show* all'interno dell'Aula e prendere voti? Io non credo sia questo Tutti i componenti della Commissione hanno presentato un emendamento con questa richiesta; e non mi si può venire a dire che è una richiesta sciocca. Tra l'altro, se il monocomponente non lo vogliono produrre le industrie farmaceutiche perché non ci guadagnano a sufficienza, facciamolo fare dall'Istituto farmaceutico militare, che è in grado di farlo.

Signor Presidente, su questo argomento ci trasciniamo stancamente. Da una parte, c'è una maggioranza che ha finanche finanche in uggia chi si pone dei problemi e chi pone dei problemi, perché deve evadere l'imperativo categorico di approvare la conversione abbiamo un Ministro che dice corbellerie come quelle che poc'anzi ha detto, ovvero che ha valenza scientifica il fatto

farmaceutico militare, che è preposto finanche a fronteggiare la guerra batteriologica e chimica. Esso, cioè, dovrebbe produrre dei vaccini o degli antidoti

perché tanto costa alla sanità, non siamo in grado di attrezzare questa istituzione, già presente e già funzionante, per fare i vaccini monodose?

È un interrogativo ininfluente in quest'Assemblea, dove abbiamo dissertato per giorni sul sesso degli angeli? Ci troviamo di fronte alla più patente delle sconfitte dello Stato che si piega alla logica mercantile di chi dice: o compri il mio prodotto, o il prodotto non te lo fornisco

con il quale abbiamo vaccinato 14 milioni di bambini italiani, dieci anni dopo il Canada e cinque anni dopo la Germania. Solo dieci anni dopo l'AIFA ha dichiarato questo vaccino portatore di complicanze e danni.

una spesa inutile, ma non c'è alcun danno. C'è soltanto un rinforzo della risposta immunitaria. Premesso questo, secondo me è buona norma indicare

adeguata all'uso, quindi monovalente per il vaccino e monodose per altri farmaci. Stiamo attenti a dire in queste istituzioni cose che non sono vere, tipo trarre conclusione di danni o alludere a motivazioni diverse da quelle che hanno

questa Assemblea e tutti i cittadini italiani devono sapere - ce ne sono a decine di migliaia che ci stanno ascoltando - che la relatrice e il Governo esprimono un parere contrario a un subemendamento

è fondato sull'antiscienza, perché non si può scrivere che se uno è immunizzato da malattia può essere esonerato

intervengo molto brevemente. Io appartengo a quell'ampia parte di Paese che ritiene i vaccini fondamentali. Ho applicato ai miei figli questo principio e, infatti, sono vaccinati su tutto, ben prima di questo decreto-legge. Ritengo che su questo punto si stia commettendo un grave errore:

nella difesa di questo decreto-legge e della salute dei cittadini, di avere solo quello come faro. Le motivazioni e le argomentazioni rispetto all'industria e alla sua organizzazione dovrebbero stare fuori da questa Assemblea, perché ci stiamo occupando di un tema delicato. Signor Ministro, non ho intenzione di fare polemica, ma ritengo ci sia bisogno di avere rispetto dei parlamentari e anche del sottoscritto, che è un ignorante in tema scientifico, ma che ha una sensibilità, che non è quella che abbiamo sentito attraverso discorsi surreali

subemendamento aggiuntivo all'articolo 5 senza

aggiuntivo all'articolo 5 senza aver votato l'articolo 5? Credo che qualche problema si ponga.

prendendo un farmaco combinato mi sottopongo a un rischio inutile e potenzialmente dannoso.

Se il farmaco monocomponente non serve nei casi in cui una persona è già immunizzata per cui lo fa solo rispetto alle malattie

la seduta va sicuramente sospesa, ma non mi si dica per cinque minuti, perché il problema non lo si risolve convincendo i riottosi della maggioranza, ma dando risposte di buon senso e accettando questo subemendamento.

La seduta è ripresa. Mi scuso con i colleghi per il ritardo con cui è reiniziata la seduta, però credo che il tempo trascorso sia stato molto utile e si sia fatto

all'emendamento 1.1500 della Commissione, avevo evidenziato - e lo ribadisco qui - quanto avessi ascoltato e recepito la preoccupazione di quest'Assemblea, che ho sentito di nuovo questa mattina in sede di discussione, rispetto a due grande temi. Il primo è quello dei cittadini e delle famiglie che vogliono tutelare e tutelarsi rispetto a una ripetizione di vaccinazione, quando immunizzati rispetto a una malattia infettiva, essendoci sul mercato a disposizione in questo momento solo formulazioni pluricomponenti. Il secondo tema era la necessità di lanciare un segnale chiaro al mercato del farmaco, all'industria farmaceutica, alla produzione del farmaco, rispetto ad interventi per la produzione di vaccini monocomponenti. Non saremmo stati in alcun caso rispettosi dei cittadini e delle loro preoccupazioni se solo avessimo scritto che si poteva fare il vaccino monocomponente sapendo che non esiste, e forse non era sufficiente la formulazione «per stimolare la produzione e la messa sul mercato dei vaccini monocomponenti».

Il comma 2 parla dell'avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale comprovata da certificazione, che esonera dall'obbligo della relativa vaccinazione. «"Conseguentemente il soggetto immunizzato adempie all'obbligo vaccinale di cui al presente articolo, di norma, con vaccini in formulazione monocomponente

«2-*bis*. Al fine di cui al precedente comma, le procedure accentrate di acquisto di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 e di cui all'articolo 1, comma 548 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con riferimento all'acquisto dei vaccini obbligatori, riguardano anche i vaccini in formulazione monocomponente».

Si riprenderà a trattare l'argomento e ciascuno potrà argomentare come voterà, ma non riapriamo la polemica inutilmente.

tutte le varie tematiche che sono state discusse in questi giorni e che erano rimaste irrisolte. Credo che la sua portata e le soluzioni che propone sia tale

credo che sia stata fatta una valutazione. Ho letto la relazione tecnica con la quale si è tentato di spiegare il subemendamento della relatrice e questa lascia numerosi dubbi, visto che comunque la relazione tecnica sul nostro emendamento e su quello della Lega non c'era mai stata (e voglio che resti agli atti). Io le chiedo

La RAI è paralizzata in mancanza di un piano di riforma che andava già attuato molto tempo fa. Ci sono i palinsesti che stanno partendo per l'autunno e non possiamo continuare a rimandare questo incontro. Anticipare l'inizio dei lavori d'Assemblea alle 15 significherebbe impedire alla Commissione di vigilanza RAI, che

Presidente, io credo che la proposta che lei ha sottoposto all'Assemblea sia del tutto condivisibile, anche perché questo è un tema eticamente eticamente e socialmente molto avvertito e credo si debba dare risposta non solo al decreto stesso e al suo percorso, ma anche a quest'Assemblea che già da diversi giorni si sta impegnando su questo tema. Quindi, a nome del mio Gruppo, ritengo di accettare pienamente e condividere la proposta che lei ha sottoposto all'Assemblea.

certamente accelerare e recuperare il tempo che stamattina abbiamo perduto, quindi siamo assolutamente d'accordo sulla proposta di riprendere i lavori

come ha detto la senatrice Taverna, noi dovremo esaminare anche i subemendamenti quindi non vorrei che poi facessimo uno *stop and go*. Se dobbiamo esaminare l'emendamento della relatrice abbiamo bisogno anche della relazione tecnica perché, essendo appunto un emendamento della relatrice, è opportuno che sia sia corredato dalla relazione tecnica; poi dobbiamo ricevere i subemendamenti; quindi io posso convocare in modo utile la Commissione quando l'intero pacchetto è pronto, altrimenti rischiamo, come tante volte succede al di là della volontà di chiunque, di dover sospendere di nuovo la seduta per fare un'altra verifica. Suggerirei un'ipotesi per la quale si fissa un termine per i subemendamenti e successivamente a tale termine si può convocare utilmente la Commissione bilancio.

La seduta è ripresa.

alcuni dei quali sono stati presentati dalla Lega

clamorosamente smentito. Inoltre, visti la preoccupazione e l'imbarazzo che si stavano palesando in Aula, è stata chiesta una sospensione

Il tema dell'immunizzazione da malattia e il conseguente esonero dall'inoculazione di quel vaccino sono stati posti dal Governo, ma appunto con dei bachi.

essere oggetto di inoculazione di un vaccino che porta in sé dei rischi. Non bisogna far quindi correre rischi inutili a un soggetto già immunizzato, perché l'inoculazione dello stesso vaccino potrebbe far registrare una sorta di iperimmunizzazione, stimolare il sistema immunitario in modo non appropriato e determinare l'insorgenza di patologie autoimmuni. Il testo del decreto-legge era stato oggetto di critiche anche da parte della Conferenza delle Regioni, che ovviamente - come detto anche da noi la scorsa settimana portato con sé dei rischi di insorgenza di numerosi contenziosi tra i cittadini e lo Stato.

dallo stesso ministro della salute Lorenzin il 21 luglio 2015. Si trattava di un'interrogazione parlamentare che toccava il tema della legge n. del 1992, recante «Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati»; una legge voluta nel 1992, che indennizzi ai soggetti che, a seguito di vaccinazioni obbligatorie, hanno riportato danni irreversibili. Ebbene, ministro Lorenzin, lei, con la risposta del 21 luglio 2015, ha affermato che alla data del 31 marzo 2015 i beneficiari dell'indennizzo aggiuntivo, in quanto riconosciuti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie,

a seguito di decesso. Quindi lei, ministro Lorenzin, con questa risposta ha messo nero su bianco la presenza di reazioni avverse

a seguito di reazioni avverse per somministrazione di vaccini. Io cito due casi:

causa ed effetto sulla morte. Cito un altro caso, riferendomi sempre a una lettera del Ministero della salute del febbraio 2011. Questa volta il suo Ministero riconosceva la morte, a seguito di vaccino, del signor Matteo, deceduto il 2 giugno 2010. Queste, Ministro, relatrice Manassero, non sono delle *fake news.* Questa non è antiscienza. Questi sono dati che avete comunicato voi, ossia lei, ministro Lorenzin,

l'emendamento della Lega Nord non ha valenza tecnico-scientifica e che gli obiettivi che il Governo si sta proponendo con il decreto-legge in esame domando, allora, di spiegarci quali sono gli obiettivi del Governo. Certamente non sono quelli del cittadino, ma sono gli interessi magari dell'industria del farmaco. Ci piacerebbe sapere che cosa ha concordato lei nel settembre 2014, al Global Health Security Agenda alla Casa Bianca, a Washington, alla presenza di Obama e del Presidente dell'Aifa. sede, ha dato la disponibilità del nostro Paese a condurre per cinque anni la strategia dei piani vaccinali nel mondo, ponendo l'obbligatorietà dei vaccini, che sicuramente ha portato al varo di questo decreto-legge illiberale. Vergogna, Ministro!

della Lega e dei vari componenti dell'Assemblea, che in maniera autonoma hanno sollevato l'obiezione sul fatto di porre un obbligo senza fornire il vaccino monovalente

multicomponenti esenti da una, due, tre o quattro patologie per l'esavalente e da una o due per il tetravalente. una discussione in Aula che si fermerà con la richiesta alla 5a Commissione di fornire una relazione tecnica che possa prevedere tutto questo, chiederei gentilmente al Ministro di riflettere qualche minuto e di essere un po' più conscia di quanto sta proponendo.

volto a sopprimere le parole «di norma» dall'emendamento 1.1600, per dare quanto meno chiarezza

viene immunizzato dalle altre malattie previste dal decreto-legge con preparati che non comprendono la malattia per la quale è immune;

legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sull'emendamento 1.1600, con la seguente condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione,

dice «nei limiti», che significa che quello che è possibile faremo e quello che non è possibile non faremo. A mio avviso, non è questo un principio corretto nei confronti dei cittadini italiani, ma non c'entrano il Presidente della Commissione e la Commissione, complessivamente, è l'emendamento creato dalla Commissione e dal ministro Lorenzin. Il ministro Lorenzin non dovrebbe giocare con il telefonino all'interno dell'Aula, ma ascoltare i componenti di questa Assemblea,

senatore Palma.

Ho sentito molte notizie che creano certamente disinformazione e allarmismi e che si allontanano dal vero nodo e dall'obiettivo che questo decreto-legge

consuetudine vuole che, se sono stato vaccinato, io possa andare a fargli visita. Qui invece viene ribaltato il problema: attenzione, sei stato vaccinato? Non ci andare.

senatore Gaetti)*. PRESIDENTE. Colleghi, ciascuno ha espresso la propria opinione e lo può fare anche il senatore Mancuso, che interviene anche di rado.

meno persone per vaccinazione che per assunzione di aspirina. *(Applausi dal Gruppo PD).* Ve lo assicuro. I farmaci hanno tutti degli effetti indesiderati, compresi i vaccini, e nella casistica degli effetti indesiderati delle vaccinazioni si va dal pianto fino alla morte

Noi riteniamo che i vaccini, efficaci e sicuri, siano uno strumento importante. Bisogna ripeterlo tutte le volte, perché c'è sempre qualcuno che tira fuori, rispetto a delle osservazioni ragionevoli che alcuni di noi fanno, l'idea che lo facciamo perché siamo a favore dei no vax. È un'altra cosa: per cortesia non tiriamo fuori tale questione. Noi abbiamo sempre preso le distanze dai no vax. Io in particolare ho preso sempre le distanze, parlo per me ovviamente ma anche per i miei colleghi.

Ci stiamo incartando su una problematica che avrebbe potuto essere risolta molto semplicemente, a mio modesto giudizio, già in Commissione sanità. questi emendamenti che propongono di prevedere la possibilità per i cittadini che avessero ragione di richiederlo, di usare il vaccino monocomponente, li abbiamo già discussi in Commissione sanità, fino alle tre

Ma io non voglio arrivare a questo punto, perché mi sembra di andare a cercare qualcosa che può essere visto come un cavillo. Dico semplicemente che bisognerebbe prevedere - lo abbiamo circoscritto a coloro che sono stati immunizzati per via naturale - che

e ce lo ripetiamo. La ragione è che il monocomponente, ancorché in molti casi abbia l'autorizzazione all'immissione in commercio, non è disponibile sul mercato perché le aziende preferiscono, ovviamente, concentrarsi sull'esavalente, sul tetravalente o sul trivalente. Qui, però, stiamo parlando dell'interesse dei cittadini, che è altra cosa. Pertanto, prevedere questa possibilità mi sembra assolutamente ragionevole mi sembra anche difficile dire che questo costa di più, perché ci sono maggiori oneri, dal momento che forse - ma non sono così sicura, avendo esaminato i dati di costo dei monocomponenti - il monocomponente costa di più della somma dei diversi componenti, ma

sia un errore macroscopico, soprattutto in questa materia in cui la gente vuole più informazione, maggiore capacità di essere presa in carico, più momenti di confronto con gli operatori della sanità e non soltanto obblighi da adempiere.

in grado di garantirli. C'è il diritto alla somministrazione e poi ci sarà anche la somministrazione con monocomponenti, però il linguaggio è lo specchio della cultura delle politiche sanitarie.

Ho ascoltato con attenzione il parere della Commissione bilancio e credo che l'apertura che, in qualche modo, la relatrice ha pensato di fare sia stata automaticamente chiusa. Infatti, prevedere che possano essere fatti vaccini monocomponente

Quindi, c'è non soltanto la tutela dei diritti di chi è stato già immunizzato da qualche malattia, ma anche il diritto di tutti i cittadini che devono vaccinarsi di scegliere la monodose. monodose. Poiché stiamo facendo questa discussione a tutela dell'interesse generale e - spero - non delle case farmaceutiche, vorrei ricordare alla Ministra che

più o meno positiva di solito vengono ignorati e sento parlare soprattutto di rapporto costo-beneficio. Sono perfettamente d'accordo sul rapporto costo-beneficio, ma poiché anche io sono un medico, prima del rapporto costo-beneficio, mi interessa il rapporto rischio-beneficio, perché il mio principio è *primum non nocere*.

Funziona in questo modo, in medicina. Ciò che mi dà da pensare è che, come personaggio politico - e io penso che anche un Ministro dovrebbe agire così - sia io che il Ministro siamo qui al servizio del nostro ruolo. Ma quando siamo di fronte a un decreto di questo tipo, sembra quasi che il nostro ruolo sia messo prima del servizio che dobbiamo dare allo Stato.

bilancio non ha parlato di disponibilità del vaccino, bensì di disponibilità economica. Il che è ancora peggio, perché noi rischiamo, anche qui, di fare la stessa cosa che abbiamo fatto con l'epatite C.

il monocomponente per altre tremila persone. Secondo quale criterio medico mi posso comportare così? Quindi, noi facciamo come abbiamo fatto

Su un sistema sanitario che ci costa, nominalmente, 110 miliardi più qualche altra miliardata di debito, noi dovremmo capire, in termini assoluti, questo maggior esborso

di pochi mesi o pochi anni. Ascoltavo prima l'accorato appello del senatore gli applausi che ne venivano perché, a quanto pare, qui chi ha perplessità, come diceva in maniera egregia la senatrice Dirindin, passa per un cavernicolo, per qualcuno che non vuole i vaccini.

ha ritirato dal commercio e posto in quarantena il vaccino riguardante il meningococco dei gruppi A,C e Y e l'oligosaccaride della difterite. Mi auguro che l'Aifa

tra qualche mese poteva essere iniettato ai nostri figli e ai nostri nipoti. C'è qualcuno che può confutarlo? Allora mettiamoci un po' con l'animo in pace.

si preoccupano di quante stringhe per le scarpe devono comprare e non di quante volte andare a cena fuori o a teatro. Manca la base non solo del buonsenso, ma della serietà. In questa discussione l'approssimazione e la tracotanza dovute all'obbligatorietà sono pari solo alla superficialità e alla furbizia con le quali si è approcciato il problema e lo si vuole portare a termine, come se fosse un compito di natura squisitamente politica. Quali subemendamenti ho proposto? Sempre quelli derivanti dal buonsenso: ho proposto, oltre all'eliminazione delle parole «di norma», che lo Stato italiano chieda per tutti i vaccini, sia per quelli monodose e monocomponente che per quelli polivalenti, che contengano solo ed esclusivamente l'antigene dell'agente patogeno batterico virale che che riguardi la vaccinazione che intendiamo praticare e non contengano assorbenti, additivi, nanoparticelle e altre sostanze che niente hanno a che vedere con l'effetto immunizzante del vaccino.

monodose, vaccini privi di sostanze, additivi, conservanti, metalli pesanti e altre schifezze, di cui sono composti attualmente i vaccini, potremmo pretendere!

Il discorso è questo ed è il contrario. Perché volete imporre al popolo italiano di vaccinarsi e volete convertirlo a colpi di vaccino sulla testa?

nel proprio organismo sostanze che con i vaccini non hanno niente a che vedere. Me la sapete dare una risposta? Ho aggiunto un altro subemendamento, secondo cui i vincitori delle gare pubbliche

Non ci si può prendere solo il filetto, ma si deve mangiare anche lo spezzatino, perché chi garantisce i filetti se n'è fatto portare qualche chilo a casa.

Questo è ciò che vi sto chiedendo e non sto dicendo che siete stralunati perché volete vaccinare i bambini. C'è la tracotanza dello Stato etico, che vuole rompere il nesso sacro del diritto naturale, che intercorre tra genitore e bambino e vuole interporre il proprio modo di vedere la tutela della salute dei ragazzi e dei bambini. tale Stato non ha la minima preoccupazione ad iniettare sostanze che non hanno niente a che vedere, con vaccini che vengono ritirati dal commercio dagli americani. Tra quanti anni lo ritireremo dal commercio e lo metteremo in quarantena, anche in Italia? C'è qualche medico o qualche scienziato qua dentro che me lo sa dire? Dove sta la farmacovigilanza? Andiamo a rimorchio degli interessi delle case farmaceutiche, perché in Italia abbiamo messo in ginocchio sia la ricerca che la farmacovigilanza.

e si dimenticano i fondamenti, non solo della ricerca scientifica, ma anche i dati scientifici. Cercherò di dare una risposta rapidissima, attraverso una bibliografia ben chiara, che è stata continuamente richiamata, ma non riportata nella sua integralità. integralità. Si è detto che più vaccini farebbero male. Secondo l'Aifa «se davvero i vaccini indebolissero o compromettessero il sistema immunitario, ci si aspetterebbe una minore risposta immunitaria in seguito alla somministrazione di più vaccini contemporaneamente rispetto alla somministrazione di un vaccino per volta, invece non è così». della senatrice Fucksia)*. «Gli studi clinici dimostrano che la somministrazione contemporanea del vaccino esavalente» insieme al vaccino «contro lo pneumococco, oltre a non determinare un aumento degli effetti collaterali severi, non produce una risposta inferiore rispetto alla somministrazione separata senatrice Fucksia)*. Per una sorta di legge del contrappasso, si tratta di una ricerca svolta da un certo Esposito, nel 2010. Lo stesso accade poi con gli altri vaccini, per cui si dà luogo ad un calendario di vaccinazioni dell'infanzia. Si è detto anche che la somministrazione di un vaccino ad

dobbiamo rispettare i cittadini e far sì che si possa prevedere una vaccinazione per singola malattia (quindi arriveremmo a circa 10 o 12 iniezioni ripetute, ma lasciamo stare),

non volevo intervenire ma credo sia giusto sottolineare anche la posizione di chi è a favore del provvedimento in esame, di chi pensa che l'Istituto superiore di sanità non sia un'associazione a delinquere di incompetenti.

il senatore Mancuso nel ricordare che qualora la persona già immune riceva una vaccinazione per la stessa patologia a mo' di richiamo, vedrà fortificarsi ulteriormente il suo sistema immunitario. Quindi non c'è alcun rischio e l'idea del sovraccarico vaccinale semplicemente non esiste è priva di fondamento scientifico. Questo è stato studiato anche da un punto di vista epidemiologico, in alcune combinazioni; si pensi ad esempio ai militari e alle

che la vendita dei vaccini rende conto - questo era un documento dell'Aifa - dell'uno per cento della spesa sanitaria nazionale. Le industrie farmaceutiche non diventano ricche grazie ai vaccini, quindi il loro lavoro è un buon investimento per noi. Quel lavoro è stato così sofisticato nel tempo ed è così migliorato che, pensate, quando ci vaccinavamo tempo fa con pochi vaccini, il nostro sistema immunitario era sollecitato da 3.000-4.000 antigeni (stimolazioni antigieniche), mentre oggi, con una manciata di vaccini, siamo sotto i 100. Per questo l'idea dell'iperstimolazione vaccinale non esiste. Concludo veramente in tutto il mondo, si va in una direzione. Non esiste Stato che abbia sviluppato il monocomponente. Ci sarà una ragione per cui anche la Gran Bretagna va verso l'esavalente?

RI))*. Signor Presidente, ha detto bene la collega Cattaneo: l'industria farmaceutica non si arricchisce con i vaccini.

per un inappropriato ricorso alla terapia antibiotica, se ci ricordassimo che ci sono delle mozioni presentate per impegnare il Governo a introdurre degli elementi di correzione nel nostro Paese, che in Europa detiene il primato del consumo degli antibiotici, probabilmente anche l'appassionato dibattito che si sta svolgendo in Aula potrebbe essere scritto dentro la pagina nobile di un confronto. Poiché ciò non avviene, questa non è una pagina nobile di confronto, ma una squallida speculazione politica. essendo immunizzato, essendo vaccinato, perché appartengo ad un Gruppo, quello di Direzione Italia, che per amore di coerenza e di lealtà ha fatto scelte chiare e granitiche, che mi porterebbero a confermare ancora una volta la nostra posizione di alternatività rispetto a quella del Partito Democratico e del Governo. riteniamo, che la buona politica sia una politica di responsabilità, che non deve trasformare il dibattito in un congresso della società italiana di immunologia o in un confronto confronto di natura scientifica. La politica deve accompagnare le acquisizioni scientifiche e deve fare in modo che divengano patrimonio per scelte oculate e responsabili, in quanto attengono i profili di tutela della salute e su questi temi non si può speculare.

che trasferisce l'impegno dall'articolo 5 all'articolo 1 rende consequenziale, corretto e coerente quanto è esposto nel comma che introduce la non obbligatorietà della vaccinazione per i soggetti che sono già immuni da una determinata patologia, ma ma bisogna fare il passo successivo, che personalmente ritengo sia realizzabile anche attraverso un atto solenne di impegno del Governo ad introdurre incentivi affinché il vaccino monocomponente possa essere realizzato da chi ha il dovere di farlo. Certamente non può farlo lo Stato, a meno che non imponga, con dotazioni finanziarie adeguate, questo tipo di attività di produzione allo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze. Sulla base di queste considerazioni, mi riservo di scendere nel merito anche

che si introducano elementi di incentivazione alla disponibilità concreta dei vaccini attraverso un apposito decreto che stabilirà le modalità perché questo avvenga, eventualmente disciplinando adeguatamente apposita attività negoziale con l'industria,

la somministrazione di vaccino a persone vaccinate ha delle differenziazioni a seconda dei vari tipi di malattia. Ho parlato anche con altri colleghi ed i lavori specifici su questo argomento non sono ben chiari.

il fatto che ormai in Italia ci sono le competenze per fare i vaccini attraverso lo Stabilimento chimico farmaceutico militare, quindi ci sono realtà italiane che sarebbe il caso di sviluppare sempre di più per renderci sempre più indipendenti. Credo che la cosa non darà fastidio a nessuno, proprio per il fatto che

«Dopo il comma 2-*bis* aggiungere il seguente: 2-*ter*: Annualmente l'AIFA pubblica sul proprio sito istituzionale i dati relativi alla disponibilità dei vaccini in formulazione monocomponente e parzialmente combinati».

sulla bontà dei vaccini, volendo suddividere quest'Assemblea tra i sì vax e i no vax. Noi non cadiamo in questo imbroglio: qui non ci sono no vax. Noi riconosciamo l'importanza dei vaccini e le conquiste che questi hanno consentito di fare nel corso dei decenni; i nostri emendamenti, l'1.91 e i subemendamenti, volevano solo sanare, lo ripeto, le lacune presenti al comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge che, come avrebbe detto Fantozzi, «è una cagata pazzesca»! Equesto è innegabile*. Presidente. Con questo subemendamento diciamo solo che, nelle more della produzione dei vaccini monocomponente, i soggetti che sono già immuni

non è un problema di maggioranza o di opposizione. Se mi permette una riflessione anche sullo stile, visto che è stato richiamato Fantozzi, io richiamo Corazzini: «Quanta di sogni ardimentosa messe nasce in un cielo e muore in un pantano!». Io citazioni non voglio farne ma al di là delle citazioni, i decreti-legge vanno convertiti o non convertiti in sessanta giorni. Poi vi arrangiate voi.

1.1500/27 (testo 2), entrambi riferiti alla formulazione monocomponente del vaccino. Risulta altresì precluso l'emendamento 1.91, concernente la stessa materia.

intervengo per un chiarimento puramente procedurale: dobbiamo quindi ritenere non più convocata la seduta del pomeriggio?

Leggiamo il contenuto dell'emendamento.

la relatrice

Aggiungere, in fine, il seguente comma: «3*-bis*. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli operatori scolastici e gli operatori sociosanitari presentano agli istituti scolastici e alle aziende sanitarie

Presidente, vorrei sottolineare come anche in questo caso si considerino i minori stranieri non accompagnati come soggetti diversi rispetto ai minori. Siccome il nostro sistema sanitario, per fortuna, non li discrimina, continuo a ritenere sbagliato discriminarli con questo tipo di emendamenti. Annuncio quindi il voto contrario su questo emendamento.

sembra assolutamente sbagliato discriminare, nell'ambito del sistema dell'istruzione, i servizi educativi per l'infanzia e la scuola dell'infanzia, proprio dopo che abbiamo approvato, con la riforma della buona scuola, un principio di messa in filiera di questo grado di scuola con le altre.

un importante momento di formazione per i ragazzi che accedono all'istruzione pubblica. Si è anche svolta una discussione in quest'Aula in base a quella delega per ampliare addirittura

se ci troviamo al cospetto di bambini vaccinati in cui l'educatore non si sia vaccinato. Ciò a meno che non vogliate allargare l'imposizione

Senatore, non c'è bisogno di usare questi toni.

genesi. Chiedo al Ministro perché si è adottato un decreto-legge? Perché siete entrati a gamba tesa? Si sta parlando - c'è anche il Ministro dell'istruzione - di aspetti invasivi all'ennesima potenza nella vita dei nostri concittadini. Avete scelto una modalità che vuole essenzialmente utilizzare il manganello della legge nei confronti dei cittadini e questa modalità è sbagliata. Stiamo entrando nel merito di aspetti educativi, etici, di sicurezza e di sanità.

trenta secondi, per dire che tutto il Movimento 5 Stelle sottoscrive questo emendamento, perché crede profondamente nella lotta contro la dispersione scolastica. E la lotta contro la dispersione scolastica parte proprio dai primi anni

Signor Presidente, io sento qui alcuni colleghi sostenere il diritto di tutti i bambini e di tutte le bambine di poter frequentare l'asilo nido e la scuola dell'infanzia. Questo provvedimento ha esattamente questo scopo: permettere a chi non può non può prendere malattie infettive, che risulterebbero letali per bambini gravemente ammalati, di poter frequentare e accedere a un nido e a una scuola dell'infanzia o anche a una scuola dell'obbligo, perché chi della senatrice Taverna)*. Questo è il grave problema che abbiamo dovuto affrontare in Emilia-Romagna, quando un bambino di un mese è morto di pertosse e quindi hanno iniziato a intervenire i Comuni e le Regioni. Voglio ricordare infine la sentenza del TAR del Friuli-Venezia Giulia del 20 gennaio, che dice con grande chiarezza che la libertà individuale deve retrocedere rispetto all'interesse pubblico di tutela della

Presidente, qui dentro la medicina sta diventando un'opinione. Allora, volevo chiarire questo punto: è vero che ci sono dei bambini che sono immunodeficienti e che quindi non possono venire a contatto con soggetti che hanno malattie infettive. D'accordo. Però in medicina - o io studio in libri totalmente diversi dai vostri - per i bambini che presentano immunodeficienza il vero problema sono gli enterobatteri gli streptococchi. Quindi coloro che hanno il mal di gola, come ce l'ho ora io, non dovrebbero andare a scuola. Poi ci sono molti bambini immunodeficienti, purtroppo, che non hanno il problema dei non vaccinati, ma sono costretti a stare a casa a studiare...

anche segnalare di ascoltare il medico, invece di riempirsi la bocca con delle argomentazioni pretestuose e ridicole. a breve di tornare proprio sull'emendamento della senatrice Puglisi - e mi fa piacere che sia presente la ministra Fedeli - perché andremo a vedere cosa fa la senatrice Puglisi del denaro che serve proprio per l'integrazione di cui tanto si riempie la bocca.

di possibilità. Vorrei anche ricordare che, se passa questo schema, si dovranno vaccinare tutti, finanche l'autista che accompagna il bambino a scuola.

che addirittura qui, oltre che sulle tante opinioni camuffate da verità scientifiche, ma che tali non sono, ci si basa addirittura sulla lettura di chissà quali bugiardini, un'evidenza né una certezza, ma solo - appunto - opinioni. Noi stiamo compiendo un atto importante che è quello di definire un'obbligatorietà per la prima parte della vita dei bambini, perché quella è la

Conseguentemente, dire che questo non può essere fatto significa modificare radicalmente un decreto-legge che - voglio ricordarlo - è stato votato dall'intero Consiglio dei Ministri, non solo da alcuni Ministri. *(Commenti dei senatori Airola e Gatti).* Presidente, con molta tranquillità vorrei consegnarle una riflessione. Tutti siamo sereni in quest'Aula e stiamo cercando il bene di tutti.

su questo provvedimento, ma adesso non posso fare a meno di intervenire perché, con la previsione del comma 3 dell'articolo 3, signor Ministro, ella stabilisce una regola che contrasta con gli articoli 9 e 34 della Costituzione. 34 della Costituzione. Io non credo che con norma ordinaria si possa impedire l'esercizio di un diritto di rango costituzionale. Io affido a lei questa mia breve osservazione, perché lei dica se è possibile, per un verso, con l'articolo 34 prevedere che la scuola è aperta a tutti e che l'istruzione è obbligatoria:

non eccedere e quindi sopprimere il comma 3.

presentazione del certificato di vaccinazione non inibisca l'accesso dei bambini da zero a sei anni al nido e alla scuola dell'infanzia. il suo ragionamento non regge. Lei vuole tutelare gli immunodepressi; avete tentato, ma è fallito clamorosamente il tentativo di far vaccinare gli operatori scolastici

i figli di coloro che frequentano le scuole elementari decidono, di fronte alla diffidenza che aumenterà in seguito a questo decreto-legge, di non far vaccinare i propri figli perché tanto, attraverso il pagamento della sanzione, potranno chiedere e ottenere

Grazie senatore non c'è tempo perché abbiamo i secondi contati. Sento la collega che ci richiama ad una sentenza che dice che il diritto soggettivo, o meglio il diritto naturale, deve soccombere rispetto all'interesse generale;

c'è. È vero che ci sono i bambini immunodepressi - e bene ha fatto il collega Maurizio Romani a dirci che sono immunodepressi per la candida, per lo streptococco*,* per il *virus* del raffreddore e che quindi dovremmo vaccinare tutti gli altri per tutto lo scibile batteriologico e virologico umano - ma c'è un'immediata considerazione da fare. Quando il popolo...

Io vi farò omaggio tra qualche settimana dei falsi certificati che a Forcella stamperanno per le vaccinazioni già avvenute e costeranno meno dei 100 euro che è la sanzione minima. *(Applausi

il problema non è quello di fare vaccinare (perché li fanno vaccinare) i bambini, ma è quello di non trovare posto all'asilo nido, sia in quello privato, con rette altissime, sia in quello pubblico, con rette altrettanto altissime (sempre che vi sia posto). Quindi il problema vero non è l'obbligo della vaccinazione, ma trovare posto all'asilo nido, cari colleghi, cosa di cui dovremmo occuparci di più*.

Signor Presidente, premetto che sono a favore delle vaccinazioni. L'emendamento 3.40 parla della presentazione della documentazione che non può essere ostativa all'accesso trasmissioni ha dichiarato che il diritto allo studio è garantito in qualsiasi ordine e grado.

per vaccinare gli operatori scolastici e sanitari anche perché non ci vorrebbe una grande copertura in quanto si potrebbe attingere al fondo per la sicurezza del lavoro. del lavoro. Comunque l'autocertificazione falsa da parte di un dipendente pubblico sarebbe perseguibile penalmente. Accetto quindi la formulazione, ma troveremo il modo di vigilare.

bambini immunodepressi che potrebbero essere contagiati dal personale sanitario, docente o non docente. Oppure forse c'è un pericolo a seconda della fonte che veicola l'agente infettivo? Lo chiedo agli illustri medici che si esprimono aulicamente come il senatore Romano. Fateci capire: se si contagia perché il bambino non è vaccinato l'immunodepresso rischia; se si contagia perché c'è l'operatore sanitario o scolastico non rischia? Allora, scusate, innanzitutto elevo la mia protesta perché il patto Molotov‑Zanda e Ribbentrop‑Romani viene

il che prevede la sicurezza degli operatori sanitari ma verso terzi, ovverosia il medico competente, in alcuni reparti dove è particolarmente a rischio la salute dei pazienti (oncologia, anestesia) può prevedere eventualmente...

alla ministra Fedeli se fosse possibile avere una conferma di questo perché, naturalmente - e anche correttamente, se lo guardiamo dal punto di vista dell'esistenza di un'emergenza sanitaria deve riguardare tutto il personale scolastico. Stiamo mettendo nero su bianco il fatto che il personale scolastico, oltre al personale socio sanitario e sanitario, a meno che non voglia fare un falso,

come senso di civiltà e perché coerente con gli obiettivi che questo decreto-legge intende perseguire.

Presidente, l'emendamento 3.49 stabilisce semplicemente che la mancata presentazione della certificazione vaccinale non costituisce in alcun modo impedimento per l'accesso alla scuola dell'obbligo.

dell'obbligo. Con questo emendamento vorremmo avere certezza, scrivendo che la scuola dell'obbligo è un diritto costituzionale garantito e che non sarà vietata ad alcuno

cento delle persone che hanno avuto il morbillo in questi ultimi anni ha più di ventisette anni. Il problema non è per i bambini. Il problema è che oramai il morbillo - faccio questo esempio - lo prendono gli adulti perché i bambini sono già vaccinati. Allora, se abbiamo veramente

contrario, rischiamo di ottenere degli effetti quasi nulli e l'effetto *boomerang* di indurre tutti coloro che hanno qualche dubbio ed esitazione ad esitare ancora di più, perché non si capisce cosa si sta facendo.

è stato già trattato nelle precedenti sedute. Noi non riusciamo a capire perché bisogna prevedere le misure in questione esclusivamente per i minori stranieri non accompagnati. ne arrivano molti in Italia ma, parimenti, arrivano anche molti minori stranieri accompagnati. Quindi, obbligo per gli uni, con diritti e doveri, e nulla per gli altri? È un emendamento di buon senso.

4.0.5 della Commissione il parere è favorevole, ma devo recepire la condizione posta dalla 5a Commissione, inserendo alla fine le seguenti parole: "La partecipazione all'Unità dì crisi è a titolo gratuito e ai componenti non sono corrisposti gettoni, compensi o altri emolumenti comunque denominati.". Il parere

dai senatori Barani e Mazzoni.

e andare avanti. Capisco che andate di fretta, perché la vostra logica è la logica dei numeri, ma sono preoccupato per la sua immagine, Presidente.

in chiaro e pubblicati, abbiamo detto che c'è un aumento di costo, ma questo non è assolutamente vero, perché la sintesi a livello nazionale tiene conto di tutti i dati e non c'è un costo in più su un'operazione e una valutazione già fatte. Mi dispiace che questa cosa non sia stata considerata

al comma 2 contenuto nel medesimo comma; ovviamente il richiamo deve intendersi riferito al comma 1.

mi piacerebbe qui far notare un aspetto, relativo a come viene finanziato un buco che in realtà è stato lasciato in virtù della legge n. 107 e di varie finanziarie, che hanno sostanzialmente tolto il denaro con cui vengono pagati i collaboratori del preside, quelli che nella tradizione immagino tutti ricorderanno come soggetti che aiutano i dirigenti scolastici. La genialata che portava la prima firma della senatrice Puglisi andava a stipendiare e giustamente anche a compensare l'attività di questi collaboratori scolastici, dei collaboratori del preside che giustamente non possono contemporaneamente svolgere le funzioni del preside e andare in classe,

usato correttamente per i percorsi di didattica. Vorrei ricordare alla ministra Fedeli che noi parliamo di denaro che dovrebbe essere usato per l'integrazione, la formazione e per tutte

Signor Presidente, mi riallaccio idealmente all'intervento della collega Mussini e chiedo sentitamente alla ministra Fedeli di ascoltarci, perché noi stiamo coprendo questo emendamento

per l'innalzamento della scolarità e per l'innalzamento del tasso di successo della scolarità. Nel decreto-legge sul Mezzogiorno abbiamo misure per la promozione del successo del tasso di scolarità e per il contrasto all'abbandono scolastico, che sono tutte tutte cose che rientrano tra le attività alle quali dovrebbe attingere anche questo fondo. Nella buona scuola abbiamo un comma in cui noi chiediamo alle scuole di fare l'educazione alla

nell'ambito delle risorse disponibili. Già era una vergogna così, e ora andiamo a togliere ancora delle risorse disponibili per l'offerta formativa all'interno delle scuole. Questo, a casa mia, significa prendere per il naso i nostri studenti, i nostri ragazzi, ai quali viene sottratta l'occasione per il proprio arricchimento e non solo, ma anche per il *life long learning*, per l'arricchimento nel corso della vita…

L'emendamento della relatrice - purtroppo nella buona fede non abbiamo chiesto subito il riconteggio, mentre lo abbiamo fatto su quello successivo più o meno sullo stesso tema - non sarebbe passato in Commissione.

espressamente destinato al finanziamento di progetti volti alla costituzione e all'aggiornamento presso le istituzioni scolastiche. Il Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa...

voterò contro questo emendamento per due ragioni fondamentali. La prima ragione è stata già detta: c'è un problema di distrazione di risorse da una finalità primaria a una finalità che certamente non corrisponde a quella per la quale quei fondi sono stati La seconda ragione è che questo emendamento si inserisce in un contesto di contenzioso aperto da anni e certamente si complica con questa disposizione. Aggiungo che i vicari, e cioè i reggenti che devono scegliere i propri sostituti,

signora Ministra, la scuola sicuramente ha bisogno di risorse, le risorse che sono state tolte con la pessima scuola e con una serie di leggi finanziarie. Ha bisogno di risorse per le supplenze, per i collaboratori del preside, ha bisogno di chiarezza e di trasparenza. Fate un provvedimento *ad hoc*, fatelo nella trasparenza e nella regolarità,

non c'è dubbio che le scuole che si troveranno a dover affrontare la ricezione dei certificati delle autodichiarazioni avranno un aggravio di lavoro amministrativo.

quel ruolo a tempo pieno in attesa che arrivi un nuovo concorso. Non c'è alcun diritto acquisito e alcun diritto che precluda nuovi concorsi o altro. Si tratta semplicemente dare la possibilità alle persone e alle segreterie scolastiche delle scuole in reggenza di poter lavorare in modo sereno.

Presidente, sentendo l'evolvere della discussione su questo emendamento, procedo al suo ritiro.

avete soppresso poc'anzi un emendamento capestro.

Avete soppresso testé questo emendamento e avete fatto bene, perché le agenzie battono la notizia che al *question time* della Camera un noto parlamentare ha detto che Napoleone ha combattuto ad Auschwitz.

Presidente, poiché prevale, molto spesso, nell'esternazione dei propri convincimenti, una preoccupante cultura del sospetto, voglio riferire alla collega Mussini e a tutti i colleghi che hanno lo stesso tipo di sentimento o di preoccupazione che questo emendamento, si approvi o non si approvi, rende possibili, di fatto, le alternative ivi contenute, previste

e anche di gravi pregiudizi che sento negli interventi di alcuni colleghi, che farebbero bene ad approfondire i testi.

è ingenerata dal fatto che vi è un ritardo nell'elaborare pratiche del passato o si prevede che vi sia un sovrappiù di lavoro, al punto da rendere necessario il trasferimento di ulteriore personale per queste pratiche,

È nelle sue facoltà.

aggiungo a quanto ha già detto il senatore Malan che a me pare che sia quantomeno inopportuno usare questo decreto-legge, che sta già creando tanti problemi, un emendamento che consente al Ministero di avere venti persone in più alle proprie dipendenze quando soprattutto non si consente ai servizi vaccinali di utilizzare neanche le risorse già destinate ai programmi di vaccinazione per assumere, ad esempio, del personale. Pertanto, se c'era un problema precedente, come ha detto esattamente il senatore Malan, di procedure arretrate, forse bisognava pensarci prima. Se non c'era urgenza,

fare passi avanti al personale della scuola, di fare passi avanti al personale del Ministero della salute in assenza di qualunque intervento in aiuto dei servizi vaccinali, mi sembra per lo meno inopportuno.

procedure finalizzate al ristoro dei soggetti che sono stati danneggiati anche dalle vaccinazioni obbligatorie (e abbiamo parlato ampiamente delle possibili reazioni avverse) oppure da emoderivati. Venti comandi per il Ministero della salute.

senatrice Taverna

esistono eccome, considerando che state anche prevedendo di stanziare quasi 1,5 milioni di euro perché probabilmente aumenteranno le pratiche riguardanti i danni da vaccino.

Questi sono quei momenti in cui alle persone che stanno fuori e che hanno dei dubbi riusciamo veramente a crearne altri.

appartenenti a questa categoria - si sono specializzati nel recupero delle spettanze dovute alle persone colpite sia dal virus dell'HIV sia dall'HCV allorquando non si conoscevano queste cose. Credo che tra vent'anni ci saranno i ricorsi per i soggetti che sono stati massicciamente colpiti da eventi avversi

e vorrei sapere se è possibile che nella replica il Ministro ci dia contezza del numero preciso delle istanze istanze giacenti al Ministero, anche perché non si capisce perché 20 unità e non 15, e non 40 o 50, perché in un contesto serio ‑ e non voglio offendere

e ringraziare i colleghi presenti in Aula perché questo emendamento - che stiamo per approvare o per bocciare - dice che i danni da vaccino ci sono.

quali sono i soggetti che potranno avere una pensione per la spasmofilia e i soggetti che potranno veder riconosciuta come patologia cronico-degenerativa invalidante la malattia di Menière. Di queste ci siamo totalmente dimenticati*.*

all'indennizzo per danno da emoderivati, trasfusioni e somministrazioni di vaccini. Dopo di che, l'equivalenza non è la stessa, tra l'insieme e una parte. Mentre, per quanto riguarda i danni da vaccini, è

e soprattutto, come ha detto la senatrice Bottici, se parliamo di un comando, vorremmo capire meglio al di là...

compatibilmente con i rispettivi Statuti e le relative norme di attuazione. Cosa vuol dire tutto questo? Stiamo di fatto pensando a un decreto-legge che ha valore in tutte le Regioni tranne in quelle a Statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e Bolzano,

Presidente, solo per dare una brevissima spiegazione: si tratta della solita clausola di salvaguardia che inseriamo in ogni legge dello Stato e non dice null'altro se non che si applicano le leggi dello Stato nel rispetto degli statuti di autonomia. Evidentemente le vaccinazioni sono obbligatorie anche nelle Province autonome di Trento e Bolzano. Si tratta solo dell'adeguamento eventuale a fini organizzativi.

finestra"). Per chi non avesse sentito bene, l'emendamento al titolo Tit.1, della Commissione, viene

in concomitanza con l'inizio della seduta e quindi prego la Presidenza di prendere atto di questa concomitanza e di fare le dovute considerazioni. Dopodiché non ho espresso nessun parere contrario.

del parere favorevole espresso dalla 1a Commissione permanente in ordine alla sussistenza dei presupposti di necessità ed urgenza del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, recante disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza SpA e di Veneto Banca SpA. L'ordine del giorno della seduta di domani è quindi integrato con la deliberazione dell'Assemblea sul predetto parere, il che rafforza le ragioni per l'anticipazione della convocazione alle ore 9.

Signora Presidente, con questo intervento di fine seduta continuo la staffetta con cui, assieme a tante senatrici e senatori, oggi ricordiamo ogni donna che viene uccisa per mano di un uomo a cui è o è stata legata da relazione amorosa. Lo faremo finché sarà necessario ricordare al Parlamento e al nostro Paese l'urgenza di arginare la violenza nei confronti delle donne. Il 14 luglio è stato un giorno particolarmente tragico: si sono avuti cinque femminicidi in quattro città italiane e un tentato femminicidio in cinque diverse città italiane. una nuova finestra"). Colleghi, capisco che state defluendo dall'emiciclo, ma il tema che sta toccando la senatrice Cantini è particolarmente serio e drammatico, quindi vi pregherei di farlo in silenzio e rapidamente oppure di ascoltare; infatti sarebbe anche giusto ascoltare quello che la senatrice Cantini ci sta dicendo, che dovrebbe toccarci profondamente. Senatrice, la

A Bari, una donna di quarantotto anni, Donatella De Bello, è stata assassinata a coltellate a seguito di una violenta lite con il suo compagno, ora sottoposto a fermo per omicidio volontario. A Montepulciano, in provincia di Siena, dunque nella mia Regione, una donna quarantacinquenne è stata uccisa a coltellate dal marito nella casa dove lei svolgeva mansioni di badante. Il quarto femminicidio è avvenuto a Dragoni, nel casertano, dove Maria Tino, di quarantanove anni, è stata uccisa dal compagno a colpi di pistola nella piazza del paese; stando alle prime indagini, la donna aveva deciso di interrompere la relazione. Il quinto femminicidio ha avuto luogo a Roma, dove un marito ha soffocato con una busta di plastica la moglie ottantunenne, Mirella Fiaccarmi, e si è poi suicidato lanciandosi dal balcone al quinto piano. Nello stesso giorno, a Cagliari, un uomo ha picchiato la fidanzata Manuela Picei, di ventisei anni, ora in coma farmacologico, poi, probabilmente credendo di averla uccisa, si è gettato da un cavalcavia.

Salgono così a 69 le donne che ricordiamo con questa staffetta, iniziata il 30 giugno 2016. al convegno sulla violenza sulle donne, ci dicono che il femminicidio è solo la punta dell'*iceberg* della violenza maschile nei confronti delle donne. In Italia sono 8,3 milioni le donne vittime di violenza psicologica, 4,5 milioni quelle che hanno subito atti sessuali degradanti o umilianti, rapporti non desiderati, abusi o molestie, tentati stupri. Il 20,2 per cento delle donne tra i sedici e i settant'anni è stata invece vittima di violenza fisica e minacce. Concludo. Riproponiamo con convinzione il nostro appello, un appello al Governo tutto, alla Sottosegretaria con delega alle pari opportunità: la cabina di regia deve monitorare l'applicazione, i pregi e i limiti della legge n. 119, che abbiamo approvato in quest'Aula nel 2013. cercare tutti insieme di dare piena e accurata attuazione al piano contro la violenza. Un appello ai *media*: si smetta di giustificare, anche solo con un linguaggio sbagliato, gli assassini e di colpevolizzare le donne. Infine un appello al Paese, agli uomini e alle donne: sì, perché c'è un lavoro da fare anche da parte di ognuno di noi, singolarmente e in famiglia, dove si formano e crescono i nostri figli maschi. L'esempio e gli insegnamenti che diamo a loro sono le basi su cui fondare un reale e generalizzato cambiamento, che produca un'inversione della casistica dei femminicidi e della violenza sulle donne. Sono state più di 120 le donne uccise nel 2016: non possiamo più accettare questa mattanza.

Signora Presidente, un invito per tutti gli italiani, un invito per i colleghi: se venite in Veneto, astenetevi dal bere acqua di falda.

Gli scienziati ci dicono che ci vorrà un secolo prima di ripristinarla. Capisco che a dire un secolo ci vuole un attimo; ma un secolo sono cento anni, quindi vuol dire che per cento anni, se non provvediamo a bonificarla (ed è praticamente impossibile, perché è in profondità), rischieremo di bere veleni. I PFAS infatti sono veleni, che una volta che entrano nel corpo, anche magari per aver bevuto solo un bicchiere d'acqua, ci rimangono per dieci anni: sono veleni che rimangono in corpo dieci anni. Ora, è vero che la Commissione sulle ecomafie riaprirà l'inchiesta per accertare le responsabilità, ma è altrettanto vero che i carabinieri del NOE affermano che queste cose si conoscevano dagli anni Quindi, per l'ennesima volta, siamo di fronte a responsabilità per le quali partirà, anzi è già partito il classico scaricabarile. Come è possibile che si sapesse che si sversavano in falda acquifera veleni mortali venti o venticinque anni fa e che non si sia ancora provveduto? Quello che è sicuro è che assistiamo, dai numeri e dalle statistiche, a un aumento della mortalità a un aumento delle malattie gravi. I nostri figli hanno in corpo livelli di PFAS trenta volte superiori rispetto ai limiti consentiti dalla legge. Queste sono le uniche certezze; per il resto, ci sono solo le recriminazioni, i dubbi e le responsabilità, sulle quali adesso la politica dovrà dare - speriamo - delle risposte e quanto meno meno dovrà consentire alla magistratura di punire i colpevoli perché, così come per il settore bancario, non abbiamo il numero sufficiente di magistrati per svolgere i processi penali e quindi arriveremo alla prescrizione; questa maledetta prescrizione che fa sì che non si ottenga giustizia in centinaia di casi, vuoi nei casi di reati bancari, vuoi, in questo caso, per reati di inquinamento ambientale. Ancora una volta, sollecito

fare prevenzione e di convertire i processi industriali e non è solo una necessità morale legata al fatto di non inquinare più, ma è anche una opportunità di *business*. I primi che produrranno in maniera ecosostenibile, infatti, avranno un enorme vantaggio economico, perché è chiaro che in tutto il mondo la fiscalità si sta trasferendo

*(M5S)*. Signora Presidente, colleghi, lo scorso 14 luglio, all'età di 99 anni, è venuto a mancare l'ex senatore Giovanni Pieraccini. Era nato a Viareggio il 25 novembre 1918. Giornalista, politico, appassionato di arte e musica, fu Ministro dei lavori pubblici per il Partito Socialista nel primo Governo Moro e anche Ministro della marina e Ministro della ricerca scientifica. Fondamentale per la sua crescita formativa e umana fu il liceo ginnasio «Carducci» di Viareggio, che lui frequentò. Una scuola che, nonostante la dittatura fascista, si distingueva per libertà, modernità e lungimiranza. Valori, questi, che hanno accompagnato la sua esistenza, tutta dedicata alla politica e alla cultura. Si avvicinò al socialismo durante la Resistenza, diventando direttore del quotidiano socialista «L'Avanti» dal 1958 al 1963. La sua carriera politica fu costantemente animata da una connessione sentimentale con il Paese ed i cittadini. Un episodio su tutti: nei giorni della straordinaria alluvione che colpì Firenze nel 1966, fu il primo esponente del Governo a recarsi sui luoghi della tragedia e a dare una testimonianza di vicinanza e conforto da parte delle istituzioni. Lasciò la politica attiva nel 1974, da fermo oppositore di quel graduale avvicinamento PCI-DC che secondo Moro e Berlinguer avrebbe dovuto condurre al compromesso storico. Da quel momento, dedicò tutto il suo tempo alla cultura. Nel 1986 fondò «Romaeuropa», dando vita al Romaeuropa Festival, ancora oggi uno dei primi dieci *festival* europei di cultura con partecipanti provenienti da molte nazioni. Grande cultore e promotore dell'arte, ha creato una vastissima rete di artisti, musicisti, letterati, anche stranieri, con i quali ha condotto molte battaglie culturali. Ha avuto rapporti stretti con grandi personalità: De Chirico e Calder

sia dal punto di vista organizzativo che promozionale, prevedendo la creazione di un unico *brand*, quello che lui sognava, perché l'Italia potesse riavere un grande punto di riferimento della cultura. Io ho il piacere di commemorarlo in quest'Aula e chiedo che almeno domani venga osservato un minuto di silenzio in suo ricordo.

Tale nave è stata noleggiata da un gruppo denominato Generazione Identitaria, che si dichiara apartitico ma usa toni e minacce

L'intento del progetto, che si chiama Defend Europe, e che coinvolge attivisti neofascisti di vari Paesi europei, sarebbe volto a bloccare «le barche dei clandestini impedendogli di toccare le coste italiane o europee fin quando la guardia costiera libica non verrà a prenderseli per riportarli riportarli indietro» - così hanno dichiarato - nonché ad esercitare una forma di controllo sull'operato delle imbarcazioni di salvataggio delle organizzazioni non governative. Quindi la C-Star si appresta ad aggiungere altri problemi alla situazione complessiva nel Mediterraneo, che certo non ha bisogno di ulteriori fattori di tensione, tra l'altro al di fuori di qualsiasi coordinamento con la Guardia costiera. Queste azioni di disturbo non meglio precisate potrebbero rappresentare infatti un grave pericolo sia per i naufraghi sia per il personale operante in mare, come segnala un appello sottoscritto da numerose associazioni della società civile, tra cui l'ARCI, la Comunità di Sant'Egidio e la Rete antirazzista. In un momento in cui si chiede proprio alle ONG di sottostare a regole ancora più severe per quanto riguarda le operazioni in mare, la nave C-Star potrebbe essere arrivata al porto di Catania per fare rifornimento e imbarcare i volontari arruolati con una campagna di tipo quasi paramilitare in diversi Paesi europei. Chiediamo dunque con urgenza al Governo di attivarsi e di riferire, per evitare che il dramma dell'immigrazione via mare nel Mediterraneo si trasformi in un'occasione per gesti provocatori di speculazione politica da parte di gruppi razzisti, xenofobi e fascisti e per non mettere ulteriormente a rischio la vita di naufraghi, migranti e degli stessi soccorritori, proprio in conseguenza di queste azioni di disturbo. Chiediamo che, qualora la C-Star risulti effettivamente ormeggiata nel porto di Catania o in altri scali italiani, essa sia sottoposta a controlli incisivi delle persone e dei materiali presenti a bordo (potrebbero anche esserci armi), e per precauzione sia messa comunque nella condizione di non prendere il largo. Ciò per evitare forme di interferenza con le missioni che l'Italia ha assunto nel delicato e strategico teatro del Mediterraneo, che arrecherebbero tra l'altro grave pregiudizio all'immagine del Paese e alla sua tradizione di civiltà e e accoglienza, e allo sforzo che di continuo tutti i nostri operatori fanno.

del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, recante disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza SpA e di Veneto Banca SpA. L'ordine del Grazie,